2.5/1, 4.1000, 4.500/1, 4.0.2000 (già 12.0.701), 4.0.2001 (già 12.0.702), 4.0.2002 (già 12.0.703),

7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20,

10.400/102, 10.0.900, 12.0.300 e 12.0.400 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza: parere non ostativo ad eccezione delle proposte 12.0.300 (limitatamente ai commi 5 e 6), 12.0.400, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/21 e 5.0.900 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 4.0.2001 sul quale il parere è di semplice contrarietà. Il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1000 (testo 2) è reso nel presupposto che: * gli oneri quantificati nella relazione tecnica siano onnicomprensivi anche delle spese di pernottamento; la copertura del provvedimento è limitata a sei mesi e, di conseguenza, l'eventuale proroga della missione dovrà essere disposta con un nuovo provvedimento legislativo; * la copertura sui fondi speciali relativamente all'accantonamento del Ministero degli esteri, come confermato dal Governo, non pregiudica la copertura di provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali».

necessaria perché la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha dimostrato che il testo così come è determinato e scritto consente l'applicazione e quindi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di fatto solo in caso di prostituzione. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2006, infatti,

Signor Presidente, nel dibattito che ha riguardato l'articolo 6 del decreto-legge si è evidenziata l'importanza della collaborazione tra il ruolo e le competenze dei Comuni e dei sindaci con i compiti in materia di pubblica sicurezza propri delle autorità statali presenti nei rispettivi territori al fine di garantire un ordinato svolgersi della vita civile nelle città. Tuttavia, per come è affrontato nelle formulazioni contenute nel decreto-legge, c'è il rischio che questa collaborazione di tipo partenariale determini sovrapposizioni e incongruenze tali da poter inficiare lo spirito e la chiarezza di una fattiva collaborazione. Perquesto l'emendamento 6.707 e il successivo 6.721 chiariscono cosa si debba intendere per sicurezza urbana, togliendo qualunque margine di ambiguità con le prerogative di chi deve assicurare la gestione dell'ordine pubblico nelle città e agevolando dovunque la minore cooperazione in termini partenariali nel rispetto della sfera delle reciproche competenze e responsabilità tra sindaci e prefetti. Sottolineo che il contenuto di questi emendamenti riflettono anche le proposte che 21 sindaci di città medie del Centro-Nord d'Italia hanno avanzato al ministro dell'interno Maroni in un incontro a Parma tenutosi la settimana scorsa. Inquesto stesso spirito, siccome la legislazione emergenziale non aiuta a rendere strutturali e ordinariamente più incisive le politiche di sicurezza nelle città, muove anche l'ordine del giorno G6.101, presentato insieme alla senatrice Incostante, al senatore Bianco e ad altri colleghi, per colmare un vuoto normativo che inquadri i rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e adegui il profilo della polizia locale ai cambiamenti intervenuti in 20 anni nelle nostre realtà urbane. Si tratta di temi su cui c'è ormai un'ampia elaborazione condivisa tra Regioni e autonomie e anche sintonia con le tecnostrutture del Ministero dell'interno, nonché con la generalità delle espressioni di rappresentanza delle polizie locali che puntano a valorizzare in luogo delle polizie municipali le polizie di comunità; comunità; temi ricompresi in disegni di legge presentati da maggioranza e opposizione proprio qui in Senato nella precedente e nell'attuale legislatura. Pertanto, in riferimento all'ordine del giorno, sollecito il Governo ad assumere un'iniziativa concorrente nel rispetto delle competenze di tipo statale.

urbana. Il primo pone l'esercizio di questo potere da parte dei sindaci nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno; il secondo prevede una norma di coordinamento rispetto alla circostanza che il sindaco, una volta emanata emanata l'ordinanza in materia di sicurezza urbana, trasmetta la suddetta ordinanza al prefetto per l'esecuzione dei provvedimenti di competenza prefettizia. Abbiamo proposto una norma di coordinamento che consente al sindaco, proprio per raccordare le varie le varie competenze esistenti in questa materia, di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che non è un'invasione della sfera di competenza prefettizia ma significa solo che il sindaco, che adotta un provvedimento relativo alla sicurezza, chiede al prefetto di porre in essere gli atti consequenziali. Poiché questi ultimi coinvolgono comunque più soggetti che siedono all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se il sindaco ne chiede la convocazione in qualche modo agevola un maggior coordinamento tra i sindaci e il prefetto. Questi sono i due emendamenti presentati. Poiché l'emendamento 6.1 viene sostanzialmente accolto negli emendamenti presentati dal Governo che pongono sotto le direttive del Ministro dell'interno l'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci e correttamente distinguono

Mi permetto di insistere sull'emendamento 6.2, proprio sotto il profilo propositivo, perché ritengo che dare al sindaco la possibilità non di convocare, ovviamente, ma di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza può rafforzare questo ruolo e credo che possa essere utile.

chiediamo un'attenzione particolare all'attività dei nostri sindaci. Con i provvedimenti sulla sicurezza abbiamo affidato ai sindaci maggiori possibilità di controllo del territorio; ma i nostri amministratori hanno anche bisogno di risorse,

Presidente, con l'ordine del giorno G6.103 intendiamo richiamare l'attenzione sull'esito dell'incontro tenutosi a Parma tra il Ministro dell'interno e molti amministratori locali di ogni parte politica, che, nella logica di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, hanno chiesto maggiori poteri

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sull'emendamento 6.733 riguarda la modifica del Testo unico attualmente in discussione, che ci conduce per taluni aspetti alla mutazione dei rapporti tra Stato ed enti locali,

federalismo peraltro condiviso da tutti gli schieramenti in campagna elettorale. C'era bisogno di questo, in quanto la criminalità che dilaga, legata spesso a doppio filo al fenomeno dell'immigrazione che ha invaso le nostre città e i nostri paesi, fa emergere la figura del sindaco,

Non può che essere così, visto che la figura del sindaco ultimamente è diretta espressione del voto dei cittadini. tutto ciò sia inevitabile in quanto sta emergendo sempre più l'assoluta necessità di individuare nella figura istituzionale del sindaco quelle prerogative che stiamo proponendo, considerato che il sindaco conosce direttamente, spesso in maniera capillare, il proprio territorio, soprattutto i propri cittadini e può intervenire con una visione spesso strategica, propria solo di chi vive e lavora nel territorio. Con questa convinzione siamo orientati ad attuare una specie di osmosi, che vede in parte rideterminare e spostare le competenze a favore del sindaco, proponendo che la figura prefettizia intervenga nel suo naturale ruolo di controllore solo ed esclusivamente nelle fattispecie in cui si evidenzia l'inerzia del sindaco o di un suo delegato nel fronteggiare i casi previsti dall'articolo 6 del Testo unico.

gli emendamenti presentati dal Governo accolgono la sostanza delle sue proposte, sia in termini di necessità di definire il concetto di sicurezza urbana, rinviando sulla questione ad un decreto del Ministro dell'interno che ovviamente non potrà

alla possibilità per le giunte comunali di graduare l'entità delle sanzioni amministrative. C'è solo una maggiore sinteticità per un verso ed una collocazione più organica per altro verso. Sugli ordini del giorno, Presidente,

in Commissione sul tema importante dell'uniformità dell'azione di sicurezza sul territorio. È chiaro che l'accordo con l'ANCI assunto dal Governo debba essere rispettato, ma non è pensabile che il sindaco possa emettere ordinanze senza nemmeno ascoltare il prefetto: ci troveremmo dinanzi ad una mancanza di uniformità dell'azione di sicurezza. Voglio ricordare infatti che l'articolo 117 della Costituzione, lettera *h)*, attribuisce allo Stato il compito della sicurezza. Apprezzo che questo sia un punto di incontro

ma il Sottosegretario converrà con me che è diverso qualitativamente: una norma di legge che definisce un concetto è diversa da un semplice rinvio ad una determinazione con decreto ministeriale del Ministero dell'interno, pur presupponendo di sentire la Conferenza Stato-Regioni. Quindi, insisto per la votazione

della maggioranza, perché il mio emendamento introduce il principio che il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, oltre che ispirarsi ai princìpi generali del diritto, deve rispettare le leggi vigenti.

in secondo luogo, trattiamo di una materia, quella della sicurezza urbana, che è un bene giuridico che deve essere tutelato dal sindaco, ma dobbiamo riconoscere anche che è un concetto privo di una sufficiente determinatezza nel nostro ordinamento giuridico. Per tale ragione inviterei il Governo a riconsiderare la sua posizione su questo mio emendamento.

quelli dei grandi centri urbani, ma anche ai Comuni con minore popolazione, che a volte hanno anche problemi di sicurezza pari se non superiori a quelli dei maggiori centri urbani. Proponiamo inoltre che non vi sia nessuna forma di condizionamento nello svolgimento di questi piani coordinati di controllo del territorio, che non vi sia nessuna forma di subordinazione delle attività di polizia giudiziaria delle polizie locali alle forze di polizia dello Stato, ma che vi sia fra di esse un coordinamento ed una collaborazione

per dirgli che non mi spingo ad affermare - come ha fatto ieri sul "Corriere della sera" l'ex ministro della difesa Martino - che l'uso dell'Esercito a fini interni è una vecchia idea di destra, che - dice l'onorevole Martino - il ministro La Russa continua a coltivare. Non mi spingo a dire questo, ma vi chiedo che da voi non vengano accuse che non corrispondono alla realtà delle nostre posizioni. Mi è sembrata una vera caduta di stile la dichiarazione del capogruppo Gasparri, che ha affermato che chi era contrario all'uso dei militari in funzione di ordine pubblico la pensa come i Casalesi e Totò Riina. Chiariamo bene i termini della questione. Vogliamo più sicurezza nelle nostre città, ma non siamo d'accordo con la vostra proposta. Ne abbiamo fatte tante di proposte, anche in questo decreto; e, come sapete, il 70 per cento di quelle in esso comprese in realtà è già contenuto nel pacchetto Amato. Quindi non potete presentarci come coloro che non si occupano della sicurezza. Evitiamo, pertanto, di ridicolizzare le posizioni di ciascuno.

trovata più per tenere il punto che per rispondere ai problemi. E non cambia la sostanza della questione principale, che è edulcorata, ma rimane. Si dice «preferibilmente carabinieri»: quanti? Per i carabinieri, poi, non era necessario un emendamento, bastava un ordine di servizio. Poi

Anche la legge che vige per le nostre Forze armate prevede che queste concorrano alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgano compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

L'emendamento comincia con quello che potrebbe sembrare un ossimoro: «Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità». Ma cosa c'è di eccezionale nella prevenzione alla criminalità? Poi prosegue: «ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato...». Quando comincerà quest'operazione? Non si sa. Quando finirà? Non si sa. Sappiamo che durerà sei mesi, rinnovabili per una volta. Mi dispiace, ma non vi sono assonanze con il provvedimento "Vespri siciliani", che è stato in qualche modo copiato per il testo. Lì la situazione era tutt'altra, dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino, era tutt'altra situazione di emergenza. Allora, è giustissimo dare risposte sulla sicurezza, ma queste risposte devono essere serie. Vi siete chiesti perché tutti i sindacati di polizia sono contrari?

questo emendamento non mi pare serva. E parlo del pattugliamento. La logica emergenziale porta all'emotività dell'opinione pubblica, ma il tema della sicurezza ha bisogno di misure strutturali, che durano nel tempo. Vi è il pericolo di trasmettere l'idea di un Paese non in grado di garantire, per via ordinaria, impegnando le forze di polizia a tale scopo preparate, la sicurezza. Puntare sulla paura può servire anche a vincere le elezioni, ma non a governare una grande democrazia occidentale.

di una norma inutile che autorizza il Ministro dell'interno, attraverso le prefetture, di concerto con il Ministro della difesa, informando preventivamente il Presidente del Consiglio e successivamente le competenti Commissioni parlamentari,

che potrebbero essere destinati, ad esempio, come ricordava nella precedente legislatura il ministro Amato, per pagare gli accasermamenti e i contratti per le prefetture, per le questure, per i Vigili del fuoco e così via, per aggiornare e ammodernare il parco mezzi della Polizia di Stato, che ha elicotteri ormai datati, che possono partecipare solo alle sfilate degli elicotteri d'epoca. Potrebbero essere utilizzati per ricominciare a discutere seriamente degli aumenti contrattuali del personale delle Forze di polizia e del comparto sicurezza. Dovrebbero essere destinati a quelle indennità che i sindacati di polizia all'unanimità chiedono e hanno chiesto al precedente Governo Prodi senza avere alcun riscontro riscontro e che chiedono ancora oggi; essi hanno presentato appositi documenti proprio perché ritengono non che siamo in Colombia, ma che questa sia una norma inutile e ancor più inutile nel momento in cui si vincola - giustamente, perché non si può fare altro - l'utilizzo di personale appartenente all'Arma dei carabinieri e che spreca risorse per fare solo uno *spot* post-elettorale. avremmo compreso e avremmo votato una norma che prevedesse l'utilizzo del personale delle Forze armate per la vigilanza non solo dei siti

utilizzasse il personale della Forze armate per la vigilanza di quelle postazioni sensibili che impiegano personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri che verrebbe liberato per compiti d'istituto. Sarebbe stato razionale, lo avremmo votato. Questo è solo uno *spot* che, obiettivamente, non fa piacere a nessuno e che, tranne la soddisfazione di un articolo sui giornali, non porterà alcun beneficio neanche alle casse dello Stato.

soldati in circostanze definite eccezionali a noi non sembra militarizzare il nostro territorio. Domandiamoci:

Voi pensate che a queste persone incontrare qualcuno con la divisa dia proprio fastidio? Pensate che le persone normali distinguano le stellette che portano i militari? i militari? Questo è un messaggio che rivolgiamo alla sinistra. Tutti noi probabilmente abbiamo sottovalutato i segnali che arrivavano dalla nostra popolazione, dai cittadini, in materia di preoccupazioni e, oltre le preoccupazioni, in materia di paura. Credo che la sinistra debba fare un profondo esame di coscienza:

e capire quali sono le problematiche e le domande della gente. Devono fare politica fuori dai palazzi, se ci riescono ancora, altrimenti la Sicilia sarà un monito. Quella è la fine che farà la sinistra se pensa che la risposta a qualsiasi domanda proveniente dal Paese

le Forze armate hanno il compito di garantire la difesa delle istituzioni, di difendere la società da minacce esterne e di concorrere al mantenimento della sicurezza interna

Si facevano, eccome, pattuglie e posti di controllo: forse ve ne siete dimenticati. Vi sono stati anche interventi infiniti in occasione di calamità naturali

«Il piano di impiego del personale delle Forze armate (...) è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza

esame. Esso consente alla polizia municipale, quando svolge attività di polizia giudiziaria, di accedere alla banca dati del Ministero dell'interno sui reati. Il decreto estende tale possibilità ai soli reati connessi al furto dei veicoli e alle contraffazioni di documenti. La polizia municipale è però spesso impegnata in attività di polizia giudiziaria

alle forze dell'ordine già operanti, faremmo sicuramente meno demagogia, ma faremmo un servizio al Paese.

Signor Presidente, colgo l'occasione per dare parere di nulla osta, già concordato con i colleghi della Commissione, sugli emendamenti 8.705 (testo 2) e 8.0.701

Grazie

affinché, dopo i successi conseguiti nella lotta alla criminalità organizzata da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine nello sgominare le cosche in tutte le Regioni - in cui si registrano grandi successi investigativi, si possa finalmente lanciare l'attacco ai patrimoni mafiosi.

casseforti della mafia), la dichiarazione di nullità di tutti gli atti di trasferimento considerati fittizi tra mafiosi, loro parenti e terzi,

aveva esaminato, preparando un lavoro che le Aule del Parlamento non ebbero mai la possibilità di portare a compimento. È un impegno che ci deve portare a comprendere che la presenza della criminalità organizzata in questo Paese è una ferita della nostra democrazia da sanare al più presto. Signor Presidente del Senato, ci ha incoraggiato ad inserire queste norme in un decreto-legge anche il discorso che lei ha voluto rivolgere all'Assemblea il giorno della sua elezione a Presidente e anche in altre occasioni pubbliche. Lo abbiamo fatto e siamo riusciti a farlo con un consenso generalizzato dell'Assemblea. Credo che tale circostanza possa costituire un fiore all'occhiello nella lotta contro la mafia, per conseguire quei successi che possono portarci verso la vittoria finale

a 10.4. La Presidenza si compiace notevolmente dell'avvenuta approvazione di questa norma

tratta infatti dell'istituzione di un'agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali. Sappiamo tutti benissimo come dal Nord al Sud dell'Italia ci siano problemi

"Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Presidente, chiedo una particolare attenzione

I testimoni di giustizia non sono i collaboratori di giustizia: si tratta di gente onesta che denuncia e che, tutto ad un tratto, viene prelevata dalla

Abbiamo un limite nell'attuale legislazione che riguarda quei testimoni di giustizia che non sono imprenditori. Con questo emendamento si prevede l'opportunità

oggettivo e obbligatorio facendolo diventare un'opportunità in più per il servizio di protezione dei testimoni che, qualora ne esistano le condizioni e non si ponga a rischio la tutela del testimone, si potrebbe comunque utilizzare

ripeto molto più sinteticamente le considerazioni già svolte in Commissione. Ho avuto l'onore di presiedere la Commissione sui programmi di protezione tra il 2001 e il 2006 e, in applicazione - per la prima volta - delle nuove norme sui testimoni di giustizia, la Commissione che presiedevo ha fatto in modo che più di un testimone di giustizia fosse avviato al lavoro anche con la pubblica amministrazione. Una norma come quella proposta (con le migliori intenzioni, che non si discutono) rischia di determinare un risultato esattamente opposto, perché rischia di irrigidire l'inserimento nel lavoro dei testimoni di giustizia che abbiano la possibilità di lavorare, in modo tale che neanche uno, poi, potrebbe essere avviato al lavoro. Sono disponibile - a nome del Governo, ovviamente - ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a proseguire questa attività positivamente iniziata, ma invito a riflettere sulla circostanza che persone oneste che hanno rischiato e che rischiano hanno necessità di assoluta riservatezza, che verrebbe necessariamente violata (ripeto, pur essendo le intenzioni totalmente diverse) dalla formulazione di questo emendamento. Solo questo motiva il parere contrario del Governo sul punto specifico. Presidente, sono veramente dispiaciuto di non poter accettare questa proposta. Ricordo al Governo che il contenuto di questo emendamento è il frutto di un lavoro della Commissione parlamentare antimafia che ha valutato tutti gli aspetti, l'ha approvato all'unanimità ed era stato proposto da un parlamentare allora dell'opposizione, oggi della maggioranza. Un lavoro meticoloso e accurato che prevede, signor Presidente, una opportunità in più, che non dà alcuna rigidità, ma che colma un vuoto esistente nell'attuale legislazione. Mi dispiace di non poter aderire, perché entrerei in contraddizione con una decisione unanime, ponderata in una relazione apprezzata della Commissione parlamentare antimafia

possono diventare testimoni di giustizia e non hanno alcun tipo di garanzia. Queste sono le cose che sono state discusse anche all'interno della Commissione antimafia e mi dispiace che il collega Vizzini sul punto non intervenga e non dica nulla.

Mi dispiace ricordare come in quest'Aula, purtroppo ripetutamente, ci siano espressioni di cordoglio quando i lavoratori muoiono sul posto di lavoro; quando però proponiamo un emendamento che interviene contro coloro che sfruttano il lavoro in maniera grave, con violazione di norme contrattuali o di legge o con trattamento personale degradante

si risponde in maniera negativa, dicendo ancora una volta che si condivide il contenuto ma si interverrà in un prossimo futuro. Èquanto avvenuto per gli emendamenti che abbiamo presentato in materia di traffico internazionale dei cittadini stranieri, dei cittadini stranieri, per tutelare le donne e i minori dalle violenze anche all'interno dell'abitazione e per interrompere il traffico internazionale criminale che sfrutta le donne per la prostituzione. Quindi, signor Presidente, prendiamo atto di questo rifiuto ripetuto di intervenire con norme in materia di sicurezza pubblica per fatti particolarmente gravi.

per dire ai colleghi - e in particolar modo al sottosegretario Mantovano - che abbiamo approfondito questi aspetti nelle Commissioni.

chiarisce un concetto ovvio, ossia che alle assunzioni si procede nei limiti delle risorse che il bilancio dello Stato e la legge finanziaria mettono a disposizione delle amministrazioni dello Stato; quindi,

un inciso secondo cui «con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate». È ovvio, infatti, che il presupposto della collaborazione del testimone di giustizia sia la segretezza, che deve essere garantita anche nell'ambito dell'accesso alla pubblica amministrazione. Poiché, però, l'articolo 97 della Costituzione prevede la riserva di legge per l'accesso ai concorsi pubblici, è chiaro che ci vuole un'esplicita deroga da parte del legislatore per consentire l'accesso alla pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia senza che ciò avvenga con un concorso pubblico. Grazie

si occupa delle strutture di assistenza ai testimoni di giustizia, si individueranno le forme più opportune per garantire la segretezza. Questo aiuta, e parecchio, soprattutto nel contrasto ad una serie di reati

Presidente, vorrei far notare, anche sull'emendamento 12.0.5, un fatto singolare. Da anni diciamo tutti che lo Stato non può pagare ai boss mafiosi, con sentenza passata in giudicato, lo strumento del gratuito patrocinio; lo diciamo da anni. L'emendamento è formulato secondo il contributo che da anni ha fornito la Commissione parlamentare antimafia; anche qui c'è stato sempre un giudizio unanime riguardo ai boss mafiosi che già hanno una sentenza passata in giudicato. Faccio un esempio: il boss Provenzano in questo momento utilizza il gratuito patrocinio nonostante abbia alle spalle delle sentenze già passate in giudicato. Il costo di questo dispendio di soldi e di questa ingiustizia raggiunge la somma di 12 milioni di euro l'anno. Esprimere un parere contrario

di fornire una risposta perché non vorrei che, come sui testimoni di giustizia, si desse un segnale così negativo, piuttosto che continuare a dare dei segnali positivi come abbiamo fatto sulle misure di prevenzione patrimoniale.

Presidente, desidero far notare all'Assemblea che, se è vero che ripugna che lo Stato paghi gli avvocati ai boss mafiosi, è altrettanto vero che si rischia di incorrere in un grave in un grave vizio di illegittimità costituzionale in questa norma perché andiamo a creare una differenziazione, nell'ambito del gratuito patrocinio, tra condannati per determinati reati e condannati per altri reati. La regola del gratuito patrocinio è che il condannato che si trovi con un reddito inferiore ad un certo limite ne possa godere. Allora il problema è di tipo diverso; non è un problema di differenziazione tra gli uni e gli altri reati, perché so perfettamente che alcuni boss mafiosi hanno patrimoni enormi, celati allo Stato, che vanno colpiti; è evidente. È altrettanto vero che la manovalanza mafiosa ha patrimonio prossimo allo zero e rientrerebbe anch'essa nella regola del gratuito patrocinio. Bisogna rivedere l'intero istituto del gratuito patrocinio, perché con questa norma si rischia di creare una disparità di trattamento e non credo che sia questo il luogo. Guarderei piuttosto ad una rivisitazione complessiva dell'istituto, perché conosco perfettamente e ripugna anche a me questo tipo di esborso che lo Stato è costretto a fare. Tuttavia, ci sono delle regole che vanno riviste con la dovuta attenzione, evitando

Sono due giorni che esaminiamo norme che violano la Costituzione; ora che si parla di mafiosi, il senatore Centaro si ricorda della Costituzione.

con una legislazione eccezionale. Per questo credo sia opportuno approvare poc'anzi abbiamo approvato un'importantissima normativa sui sequestri, che nasceva da un emendamento presentato dai relatori. Credo che sulla normativa antimafia in quest'Aula ed anche in Commissione non vi siano stati steccati. È positivo registrare questo clima. *(Applausi).*

che i magistrati potrebbero, con un'applicazione meno burocratica della norma e un'interpretazione più ad ampio respiro delle norme esistenti nell'ordinamento, disvelare, anche in via di presunzione, i patrimoni di cui dicevo e quindi negare il gratuito patrocinio. Tuttavia, detto questo - non me ne voglia il senatore Garraffa - credo che il Senato non debba

che nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, particolarmente esposti, si istituiscano sezioni dirette da presidenti di sezione, che servono non ad aggravare l'attività giudiziaria, ma a renderla più tranquilla, più serena e più garantista. A questo serve istituire i presidenti di sezione, che devono decidere anche sulla libertà delle persone. Alla lettera *c)* si prevede che nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi Regioni molto esposte, si istituiscano posti di procuratore aggiunto, nel rapporto previsto dalla legge. Spiegatemi perché vi

Grazie

come immagino farà fra qualche minuto, intende ritirare l'emendamento 5.0.900 che ci era stato sottoposto. Per questa ragione non abbiamo espresso il nostro parere.

Presidente, prendo atto con grande rammarico che il Governo intende ritirare questo emendamento, utile e necessario al disegno complessivo al fine di rafforzare la presenza della magistratura nelle sedi disagiate. Mi auguro davvero che quanto ascoltato in quest'Aula corrisponda ad un intendimento

ex volontari in ferma breve che, essendo rientrati nella graduatoria degli idonei per entrare nell'Arma dei carabinieri, come previsto dal bando sulla base del quale erano stati reclutati, si trovano ora fuori dall'Esercito e fuori dall'Arma dei carabinieri, perché il precedente Governo li aveva fatti uscire dall'Esercito in attesa di chiamarli nell'Arma dei carabinieri. Il risultato è che ci sono 224 persone, molte delle quali capifamiglia,